ringrazio la senatrice interrogante per avere chiesto al Governo chiarimenti in ordine ai rapporti tra le previsioni della contrattazione collettiva e le disposizioni normative in materia di congedo parentale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 105 del 2022. Il Governo è particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con riferimento alla doverosa conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze delle famiglie. In questo contesto il sistema delle tutele apprestate dai cosiddetti congedi parentali ha conosciuto un'importante novella con l'adozione del decreto legislativo n. 105 del 2022, emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. L'articolo 2 del decreto ha previsto che «i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva». La *ratio* della norma è quella di parificare, sul versante previdenziale i periodi di congedo parentale all'attività lavorativa, non penalizzando quindi le lavoratici e i lavoratori che si debbono assentare dal lavoro per dedicarsi alle proprie esigenze familiari. dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la fruizione del congedo parentale non penalizzerà più le lavoratrici e i lavoratori, eccezion fatta per la fruizione dei cosiddetti emolumenti accessori, che vengono corrisposti soltanto se vi sia un'effettiva presenza in servizio, a meno che la contrattazione collettiva non disponga diversamente. Questa previsione è riconducibile a un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, secondo cui la contrattazione collettiva può derogare solo *in melius* a quanto stabilito dalle disposizioni normative. In risposta dunque al quesito posto, posso dire che nessun contratto collettivo può disporre legittimamente trattamenti inferiori alle previsioni di legge che prevalgono sempre sulle eventuali diverse disposizioni contrattuali peggiorative, non rilevando la data di stipulazione del contratto collettivo. Grazie sono soddisfatta della risposta, che rientra proprio nell'ottica in cui ci poniamo come Gruppo Fratelli d'Italia, ossia quella di rimettere al centro la natalità e prevedere di introdurre tutti quegli strumenti e quelle facilitazioni

Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, in merito al ritardo nelle tempistiche dei pagamenti agli esercenti in relazione all'utilizzo della Carta del docente, occorre preliminarmente rammentare che il Ministero, con un'apposita convenzione, ha affidato alla Consap la gestione dei rimborsi dei buoni in favore degli esercenti tramite una piattaforma per la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'amministrazione di Stato. Ebbene, il ritardo segnalato dagli interroganti si deve alla circostanza per la quale si è reso necessario avviare la procedura per il rinnovo della citata convenzione, con una validità per il triennio 2023-2025 venuto ormai a scadenza. La riattivazione della richiamata procedura di stipula ha comportato l'esigenza di attendere l'approvazione del disciplinare da parte degli organi di controllo competenti. Giova precisare che, nonostante la scadenza della precedente convenzione, il Ministero ha sempre assicurato la continuità del servizio per la gestione della Carta del docente per la relativa liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercenti accreditati. A ciò aggiungo che è intervenuta la circolare del Ministero dell'economia e avente ad oggetto la chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2022, in attuazione delle disposizioni in materia contabile. Tale circolare individuava, quale termine per la chiusura dell'esercizio 2022 per quanto concerneva l'emissione dei titoli di spesa, il 16 dicembre 2022 e, quale data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario, il 9 gennaio 2023. Le circostanze sopra illustrate e l'esigenza di integrazione documentale da parte degli organi di controllo hanno comportato dunque ritardi nell'assegnazione delle risorse da parte del Ministero alla Consap. Tuttavia, a fine febbraio, il Ministero ha avviato a favore di Consap ordini di pagamento per complessivi 83,4 milioni di euro, che attualmente sono in corso di erogazione. Tali somme saranno accreditate alla Consap secondo i termini previsti dalla necessaria attività amministrativa di controllo. Pertanto, posso rassicurare sul fatto che tutte le iniziative tese a rendere disponibili i pagamenti a Consap sono state già adottate nel rispetto delle norme contabili vigenti e che, dunque, non si ritengono necessarie ulteriori iniziative per assicurare un tempestivo flusso dei pagamenti a beneficio degli esercenti che sono, infatti, tornati ad essere erogati con le consuete cadenze regolari.

anche un settore economico importante del nostro Paese che è in generale quello della produzione culturale, perché sappiamo che non è legato solo all'acquisto di libri, ma anche a spettacoli e a una serie di attività che i docenti possono svolgere.

sugli importi bloccati. Ho ascoltato con attenzione la sua risposta: da un lato so che vi siete attivati, ma dall'altro non sono pienamente soddisfatta. Mi auguro che questo significhi veramente che nel 2023

sul tema dell'editoria scolastica, che mette fortemente in sofferenza i librai per una tensione sui prezzi non dovuta a speculazioni, ma a un oggettivo aumento del costo delle materie prime, in particolare della carta, e all'inflazione.

Grazie

approfondite nel corso di diverse riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svolte presso la prefettura di Venezia e sono strutturate in due macroaree di intervento: la prima è indirizzata al progressivo aumento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, la seconda ha come obiettivo l'attivazione di specifiche misure nel quadro delle politiche sociali adottate dal Comune di Venezia. In tale contesto, è stato anche istituito, presso il commissariato di pubblica sicurezza di Mestre, un tavolo tecnico permanente interforze che si riunisce settimanalmente con la partecipazione del Comune di Venezia al fine di coordinare gli interventi, mettendo a fattor comune le diverse competenze, e al fine di programmare azioni sul territorio anche con il supporto dei servizi Dal punto di vista strettamente operativo segnalo che le Forze dell'ordine e la Polizia locale, con l'ausilio del personale del 4° Battaglione Carabinieri Veneto, nonché dei nuclei cinofili, dei Carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Venezia e del NAS di Treviso, hanno potenziato le attività di controllo volte a prevenire le attività di spaccio di sostanze stupefacenti, riservando al contempo attenzione al contrasto contrasto dei reati di tipo predatorio. Sono stati rafforzati anche i controlli preventivi sui quartieri cittadini, mediante l'impiego della stazione mobile dei Carabinieri. Sempre sulla scorta di quanto emerso nel corso dei comitati provinciali, già a partire dalla fine dello scorso settembre sono stati disposti servizi straordinari di controllo del territorio cosiddetti ad alto impatto, con l'impiego di personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, coadiuvati da Guardia di finanza, Polizia locale, Ispettorato del lavoro e unità sociosanitarie locali. Dal 1° gennaio di quest'anno è entrato in vigore, in via sperimentale e proprio nell'ottica di massimizzare l'efficacia dei servizi di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità nell'area di Mestre-Via Piave, il nuovo piano coordinato di controllo del territorio, che ha comportato una maggiore concentrazione degli equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nella zona, con un raddoppio degli equipaggi secondo criteri di rotazione. Tale piano sta dando buoni risultati, in quanto, da un esame svolto recentemente, è emersa una complessiva riduzione del numero di interventi, specie per quanto riguarda i furti in appartamento e nei negozi. In ogni caso, ovviamente, saranno valutate eventuali altre misure che si rendessero necessarie, in accordo con le altre amministrazioni interessate. Quanto agli organici delle Forze di polizia, rammento che nell'area di Mestre l'Arma dei carabinieri è dotata di una compagnia e di una stazione, con una forza effettiva di 77 unità, il Corpo della guardia di finanza è presente con il comando provinciale e il nucleo di polizia economica e finanziaria, con una forza effettiva di 320 unità. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, il commissariato di Mestre ha un organico di 67 unità, mentre la sezione di Polizia ferroviaria di Mestre dispone di 36 unità. Quanto alle azioni positive volte a prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, il Ministero della salute, interpellato sulla tematica, ha riferito che le Regioni, in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, hanno completato la prescritta pianificazione dei piani regionali di prevenzione. Lo stesso Dicastero ha puntualizzato che nel luglio 2021 è stato istituito istituito un tavolo di lavoro interistituzionale con la finalità di definire percorsi integrati e uniformi sul territorio nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze, per la riduzione del danno e per la limitazione dei rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali. I lavori del predetto tavolo sono volti all'elaborazione di apposite linee di indirizzo per l'individuazione precoce delle persone che presentano comportamenti a rischio di dipendenza patologica con o senza sostanza. Sempre in un'ottica di promozione di azioni volte a contrastare i fenomeni delle dipendenze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anch'esso interpellato sulla tematica, ha da parte sua segnalato le opportunità offerte dal fondo istituito con la legge di bilancio per il 2022, con una dotazione finanziaria pari a due milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. L'impegno del Governo è volto a garantire un ampliamento degli organici delle Forze di polizia. Al riguardo, mi preme evidenziare che un importante e concreto risultato è già stato ottenuto con l'ultima legge di bilancio, con la quale è stato istituito, presso il Ministero dell'economia finanze, un fondo per le assunzioni delle Forze di polizia e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso, di 95 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori somme che saranno progressivamente incrementate negli anni, fino a superare i 125 milioni annui a decorrere dal 2033. **Saluto

Signor Presidente, prendo atto della risposta che è stata data dal rappresentante del Governo, che mi pare tenga conto di una situazione che necessita di un ampio raggio di interventi, che in parte si stanno facendo e che in parte devono essere compiuti. Colgo anzitutto l'occasione per ringraziare le Forze dell'ordine, che stanno facendo un lavoro molto prezioso e molto importante, sia per il controllo che per la prevenzione e per il necessario lavoro di *intelligence*. Penso che Penso che sia necessario intervenire molto anche sul fronte delle politiche sociali, dei servizi e del recupero dei più fragili. La mia interrogazione, signor Sottosegretario, è del 16 novembre ultimo scorso; come lei ha detto, il tema è presente da anni. Il 24 febbraio si è tenuta una importantissima manifestazione a Mestre, indetta da comitati e associazioni di cittadini, che ha posto all'attenzione nazionale le problematiche relative alla sicurezza e che ha soprattutto chiesto tre cose: il potenziamento e un maggiore coordinamento delle Forze dell'ordine, di cui ella ha parlato, che esercitano il controllo del territorio; il rafforzamento dei servizi per l'assistenza dei soggetti più fragili e una serie di politiche di carattere urbano, rigenerativo, che riguardano il patrimonio abitativo e che riguardano il sostegno alle attività commerciali, culturali e ricreative.

legato solo alle misure giuste che devono essere prese sulla sicurezza, ma è necessario fare anche tutta questa serie di interventi.

è bene che vengano indirizzati a politiche precise, con il coinvolgimento, oltre che del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Comune di Venezia e della Regione Veneto, per avere delle politiche che possano essere davvero efficaci. efficaci. Serve riqualificare le zone più compromesse; serve aiutare i residenti e gli operatori a sentirsi normalmente più sicuri e servono una serie di interventi che vanno dal potenziamento dell'illuminazione, alla viabilità, al pattugliamento: tutte misure che aiutano le persone a non sentirsi abbandonate. Quindi, un'azione complessiva, che io credo vada fatta anche con il coinvolgimento delle scuole, consolidando il progetto del Ministero dell'interno relativo al progetto «Scuole sicure» e coinvolgendo anche i cittadini e le associazioni. Sarebbe importante da questo punto di vista, che il Comitato per l'ordine pubblico coinvolgesse in queste politiche anche i rappresentanti dei comitati e delle associazioni

sul tema di Mestre e della sua sicurezza in termini di ordine pubblico e non solo. Per quanto ci riguarda, come Gruppo parlamentare, continueremo a mantenere viva la questione e a portarla sempre sotto i riflettori nazionali nella sua accezione più ampia, in una logica che possa determinare questo coordinamento di politiche di sicurezza, sociali, di prevenzione, legate anche alla riqualificazione del territorio. Concludo dicendo che questo tavolo sarebbe utile anche per verificare la realizzazione degli interventi legati al PNRR, riguardanti anche la città di Mestre e che dovrebbero avere il senso anche di un rilancio e di una modernizzazione del tessuto urbano e cittadino.

Signor Presidente, il personale del Corpo di polizia penitenziaria ammonta a 36.126 unità. Una presenza a pieno organico della Polizia penitenziaria costituisce inevitabilmente una ragione di maggiore tutela per i detenuti e per il personale in servizio negli istituti penitenziari, oltre che per la comunità nazionale. Per tale ragione, si procederà all'assunzione straordinaria di 1.000 unità di appartenenti al Corpo, distribuiti nei quattro anni, cui bisogna aggiungere i 1.479 agenti che a luglio prenderanno servizio terminato il corso di formazione i 1.758 agenti che, al termine delle procedure concorsuali, partiranno per il corso di formazione e raggiungeranno gli istituti entro fine 2023. Da ultimo, vi è il nuovo bando di concorso per 1.713 agenti di Polizia penitenziaria, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 8 marzo. Pertanto, entro il primo semestre 2024 saranno operativi 5.450 nuovi agenti di Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda gli attuali numeri, nel carcere di Noto il personale presente è pari attualmente a 73 unità, inferiore di 15 rispetto alla dotazione organica prevista in numero di 88 unità. Nel carcere di Augusta il personale presente è pari attualmente a 184 unità, inferiore di 67 rispetto alla dotazione organica prevista in numero di 251. personale presente nel carcere di Siracusa è pari attualmente a 237 unità, inferiore di 13 rispetto alla dotazione organica prevista in numero di 250. Quanto alle presenze detentive, presso la casa di reclusione di Noto, alla data del 7 febbraio 2023, erano presenti un totale di 151 detenuti a fronte di una capienza di 176 posti disponibili, rilevandosi una percentuale quindi di affollamento pari all'85,50 per cento. Presso la casa circondariale di Siracusa, alla stessa data, erano presenti 622 detenuti a fronte di una capienza capienza regolamentare pari a complessivi 545 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari a 114,34. Infine, presso la casa di reclusione di Augusta, sono presenti un totale di 481 detenuti a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi 364 posti, di cui 26 non disponibili a vario titolo, rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari a 142,31 Più in generale, presso gli istituti di pena di competenza del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia, alla data del 7 febbraio 2023, erano presenti un totale di 6.100 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 6.500, di cui 553 non disponibili a vario titolo, rilevandosi un indice percentuale medio di affollamento pari a 102,57 Dall'analisi di tale dato non si denota un sovraffollamento comparabile a quello che si registra in altri distretti, tanto che dal 1° giugno 2022 al 4 febbraio 2023 la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento non ha disposto provvedimenti di sfollamento di detenuti dai tre su indicati istituti penitenziari. In ordine alle carenze strutturali va premesso che, sulla base delle risorse finanziarie e professionali disponibili, il DAP non ha mai smesso di pianificare e realizzare i lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria o straordinaria necessari al mantenimento e al recupero dei compendi immobiliari. Ciò precisato, con riferimento ai lavori e ai procedimenti avviati o programmati al fine di migliorare le condizioni strutturali e igieniche degli istituti penitenziari di Augusta e Noto, si rappresenta quanto segue.

Relativamente alla casa di reclusione di Augusta, si ritiene utile premettere che nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria 2022 a cura del DAP, era previsto l'adeguamento di 10 sezioni detentive per un importo stimato di circa 5 milioni di euro. Sono attualmente in corso le attività di analisi della vulnerabilità sismica delle strutture quelle finalizzate alla redazione della diagnosi energetica, con emissione del relativo attestato di prestazione energetica. Sulla base delle risultanze di tali analisi e diagnosi sarà poi avviata la fase della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico delle strutture, unitamente ovviamente all'adeguamento dei reparti detentivi. Si auspica di poter concludere l'attività di progettazione ed avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori entro il 2023. Relativamente alle carenze segnalate in merito agli impianti elettrici, si comunica che il competente provveditorato regionale ha previsto, per l'anno in corso, un intervento di rifacimento dei quadri elettrici dell'intero istituto, per l'affidamento del quale questo dipartimento ha già confermato di poter assicurare la copertura finanziaria occorrente, stimata in circa due milioni Per quanto concerne invece la casa di reclusione di Noto, si riferisce che agli atti del competente ufficio, direzione generale di beni e servizi, non risultano segnalazioni recenti di attività e criticità rilevate, tali da dover richiedere il coinvolgimento e l'intervento diretto di questa amministrazione, fatte salve comunque le assegnazioni di fondi, assicurate già nel corso del 2021, per l'ultimazione dei lavori per recupero e copertura sotto corpo di fabbrica, destinato alle sezioni detentive e per il ripristino dell'impianto antincendio. Va infine segnalato - e merita di essere evidenziato - che i finanziamenti derivanti dall'ultima legge di bilancio vedono stanziati per il DAP, per l'anno 2023, 53 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso. Si segnalano in particolare molte risorse aggiuntive: l'incremento di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno in corso, relativamente alle misure per favorire le attività lavorative dei detenuti; 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno dei successivi anni, 2024 e 2025, destinati al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento di detenuti e condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi in collaborazione con le istituzioni coinvolte, come le scuole e le università, nonché soggetti associativi del terzo settore. Concludo con una riflessione che abbiamo già avuto modo di fare proprio in quest'Aula. Alla luce di quanto detto, ritengo che un vero recupero dei detenuti, utile per affrontare tutti i temi, anche quello relativo al sovraffollamento,

in relazione al singolo detenuto, in relazione ad un clima fruttuoso e di collaborazione all'interno degli istituti tra detenuti e personale operante e un utile vantaggio anche in relazione all'intera comunità esterna, perché il 98 per cento di chi partecipa a un programma di recupero, lavorando, esce dai circuiti criminali.

per il tramite di una incisiva semplificazione anche dell'accesso degli imprenditori alle agevolazioni previste. Con questo si potrà condurre una gestione trattamentale della popolazione carceraria più efficiente e certamente più capace di raggiungere i

prendo atto con soddisfazione di tutta la parte, contenuta nella sua ampia risposta all'altrettanto ampia interrogazione di una serie di colleghi, oltre al sottoscritto, che precisa alcuni dati che avevamo difficoltà a reperire, soprattutto rispetto a queste tre condizioni carcerarie della Provincia di Siracusa. Controlleremo tutti insieme gli sviluppi relativi ai nuovi investimenti, a quelli che sono stati già programmati e soprattutto alle assunzioni di nuovo personale, perché come lei sa - siamo in una situazione complessiva nazionale che vede un *deficit* di circa 5.000 unità. Quindi, mi sembra che con lo scaglionamento che lei ha citato dovremmo provare, se non altro, a coprire questo *gap*. Dopodiché, c'è un altro tema che abbiamo evidenziato e che rappresenta più un tema di programmazione, che non è soltanto dato dal rapporto fra unità impiegate e numero di detenuti, ma è dato dalla programmazione del carico di lavoro orario e in particolare da un fenomeno che è abbastanza diffuso e che si osserva almeno nelle carceri che noi abbiamo visitato. Mi riferisco alle

C'è un altro elemento che sfugge alle statistiche, del quale ci siamo resi conto andando proprio a visitare le carceri. Mi riferisco alla caratteristica fisica, di architettura di molti di questi edifici, che si sviluppano ovviamente in verticale, dove c'è bisogno di forme continue di controlli, assistenza e vicinanza ai detenuti, per cui non è possibile realizzare strutture nelle quali ci sono molte scale e spesso ascensori che non funzionano, dove le stesse persone devono essere presenti in più piani contemporaneamente. Ecco, questo fa sì che, da una parte, ci sia un ridotto controllo, dall'altra, anche che ci siano fenomeni che sfuggono a forme di assistenza. Un secondo evento che citiamo concerne la preoccupante crescita e incidenza di fenomeni suicidari sia presso i detenuti, specie quelli più giovani, sia presso la stessa Polizia penitenziaria, segno forse non possiamo dirlo con certezza, ma è un elemento da indagare - di un malessere complessivo, di un certo carico di lavoro, di una pressione che interessa sia queste persone sia i loro familiari, come abbiamo potuto constatare. Questo ha a che fare anche con l'altro pezzo della storia, cioè la presenza degli educatori, la parte delle attività "libere" dentro la prigione, così come tutta la parte relativa all'assistenza psicologica. Questo è un elemento che molti ci hanno segnalato, che ha bisogno anch'esso di ulteriori forme di programmazione e di collegamento con le ASP e tutta la parte di programmazione sanitaria, in questo caso regionale. Nel complesso, concordiamo ovviamente sulla parte relativa all'integrazione con il mondo del lavoro; in questo senso, in particolare una delle carceri che abbiamo citato è molto attiva da sempre in queste attività, e anzi, in un certo senso rappresenta un fiore all'occhiello da questo punto di vista; ma anche in quel carcere si lamentava la circostanza di non riuscire ad avere un numero sufficiente di persone che possono essere presenti essere presenti per piano. Quello che possiamo chiedere ulteriormente, nell'applicazione delle politiche, è di guardare non soltanto alla numerazione complessiva, ma anche alla circostanza specifica di ciascuna struttura carceraria, di evidenziare anche il rapporto di controllo che ci può essere in relazione allo sviluppo architettonico della situazione carceraria medesima, ma soprattutto di insistere sulla parte relativa all'assistenza sanitaria, in particolare di supporto psicologico, e quindi di turnazione da parte della Polizia penitenziaria. Penso che questo possa servire a migliorare lo stato complessivo di salute ed i comportamenti di tutte le persone che, a vario titolo, si trovano a vivere in questo sottomondo sottomondo chiuso, che è quello delle nostre carceri.

alle quali risponderanno il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Per questo Governo e per questa maggioranza di centrodestra gli interventi contro il caro bollette sono una priorità, come abbiamo evidenziato nella manovra economica, in cui abbiamo stanziato oltre 21 miliardi a favore di cittadini, famiglie ed imprese, proprio contro il caro energia.

grazie all'impegno di questo Governo, l'Italia è riuscita ad ottenere a Bruxelles il traguardo del tetto europeo al prezzo del gas, i cui effetti sono stati subito tangibili. Nelle ultime settimane, infatti, le quotazioni del gas sono letteralmente crollate (40-45 euro al megawattora rispetto ai 140-150 di gennaio e ai 342 dell'agosto dell'agosto del 2022). Secondo uno studio della CGIA di Mestre due terzi degli aumenti delle bollette di luce e gas gravano sulle imprese, mentre la parte restante grava sempre secondo tale ricerca, nel 2022 i rincari energetici hanno pesato maggiormente sulle tasche dei nuclei familiari meno abbienti e soprattutto sulle Regioni, in modo particolare quelle del Nord (dal Veneto alla Lombardia, all'Emilia Romagna), che sono maggiormente interessate dalla presenza delle attività economiche. Le criticità legate ai rincari delle bollette di luce e gas, seppur in un contesto di minor gravità rispetto allo scorso anno, continuano a perdurare, colpendo soprattutto, come dicevo anche prima, le famiglie coi redditi più bassi e le imprese. Purtroppo, com'è noto, è imminente la scadenza delle misure in materia di energia adottate dal Governo per il primo trimestre 2023. Siamo consapevoli che non è possibile abbassare la guardia. Proprio per questo chiediamo al Governo quali azioni intenda adottare per fronteggiare il caro energia e con quali misure intenda intervenire per continuare a prevedere forme di sostegno mirate a tutela delle famiglie più bisognose e delle imprese maggiormente esposte alle difficoltà connesse all'inflazione e ai rincari delle bollette di luce e gas.

con riferimento ai quesiti posti rappresento che il Governo, consapevole del perdurare, seppur in misura attenuata, delle emergenze legate al costo dell'energia elettrica e del gas e dell'imminente scadenza delle precedenti misure, ha allo studio un provvedimento d'urgenza. Le misure allo studio, che devono tener conto delle risorse attualmente disponibili, avranno una durata temporale differenziata, anche in attesa del nuovo quadro economico che emergerà dal Documento di economia e finanza, del perfezionamento del dibattito relativo al RePower EU

Considerato che i rincari energetici colpiscono in particolar modo le famiglie a basso reddito, il Governo intende dare maggiore certezza alla gestione dei bilanci familiari dei soggetti più deboli, riproponendo il prossimo trimestre la misura del *bonus* sociale elettrico e gas per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico con ISEE fino a 15.000 euro. Il *bonus* sociale coinvolge una platea di oltre 4,5 milioni di famiglie. È inoltre allo studio una misura che decorrerà dal 1° ottobre, con l'inizio dell'anno termico. Tale misura consisterà in un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento, che sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica. Il Governo intende poi confermare anche per il secondo trimestre 2023 la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul gas metano al 22 per cento in base alla tipologia del cliente) usato per la combustione per uso civile e industriale e prevedere adeguate misure per la somministrazione di energia termica in esecuzione di contratti di servizio di energia, nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento. Infine, il Governo sta completando la definizione di misure strutturali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Nelle more di tale riforma, per il prossimo trimestre è al vaglio un'ipotesi di rimodulazione delle misure già riconosciute per il primo trimestre sotto forma di crediti d'imposta, che tenga conto dei livelli di prezzo dell'energia del gas che si sono registrati negli ultimi periodi.

e delle finanze* - Premesso che: l'Ufficio parlamentare di bilancio nella nota sulla congiuntura di febbraio, in cui aggiorna le previsioni per il biennio 2023-2024, avverte che lo scenario macroeconomico dell'economia italiana è "circondato da un'incertezza ancora molto ampia"; Nel quadro delineato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, la crescita dell'economia è confermata per quest'anno in rallentamento, vale a dire allo 0,6 per cento, a fronte del 3,9 del 2022, mentre è previsto nel 2024 un lieve rialzo, tenendo conto però che ciò è ipotizzabile solo in presenza di un progressivo miglioramento del contesto geopolitico a livello economico internazionale. Si tratta di una stima in linea con quella del Governo, ma non con quella della NADEF che, ad esempio, prevede nel 2024 una crescita dell'1,9 Il calo inoltre - avverte sempre l'Ufficio parlamentare di bilancio - è dovuto alle componenti più volatili, soprattutto quelle energetiche, mentre l'inflazione di fondo continua ad aumentare. Questo comporta che la dinamica dei prezzi resti molto alta, più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, con la conseguenza di una forte erosione del potere d'acquisto, tutta a discapito dei lavoratori e delle lavoratrici. Più di quattro italiani su non sono riusciti a risparmiare nell'ultimo anno, schiacciati dal peso delle bollette e dal rincaro dei generi alimentari. Nel 2022 l'inflazione si è attestata all'8,7 per che non toccava fin dal 1985. I salari sono rimasti stagnanti: ad esempio, l'ultimo dato Istat dice che sono cresciuti dell'1,1 per cento; la differenza è di 7,06 punti percentuali.

fenomeno conduce al fatto che i consumi delle famiglie verranno finanziati soprattutto dai risparmi. La spesa degli italiani, che è cresciuta del 4 per cento nel 2022, nella media del 2023 dovrebbe crescere di un punto percentuale. percentuale. Come detto, la ripercussione di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza come la guerra e anche i rischi legati all'attuazione del PNRR, comporta l'erosione del potere d'acquisto degli stipendi e pone in una condizione di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto dei ceti medio-bassi. Si chiede pertanto quale iniziativa urgente il Ministro e il Governo intendano adottare per contrastare la perdita del potere d'acquisto di salari e stipendi e, in particolare, se non ritengano opportuno introdurre normativamente un meccanismo similare a quello introdotto, ad esempio, nella contrattazione dei metalmeccanici nell'ultimo contratto,

senatore Magni, in questi giorni il Governo sta elaborando il quadro di previsione macro-finanziario che sarà contenuto nel Documento di economia e di finanza di prossima presentazione. I primi dati disponibili sull'andamento dell'economia nazionale per l'anno in corso evidenziano tendenze positive che, pur in un contesto ancora caratterizzato da incertezza, lasciano ritenere che gli obiettivi stabiliti dalla Nota di aggiornamento al DEF dello scorso autunno potrebbero essere raggiunti, se non superati. Gli elevati e persistenti livelli di inflazione che hanno caratterizzato finora il quadro economico hanno colpito in misura asimmetrica le famiglie, incidendo in misura relativamente maggiore sui nuclei più deboli. Il Governo, già a partire dalla legge di bilancio per il 2023, ha confermato l'impegno a proteggere i nuclei familiari più esposti, estendendo al primo trimestre dell'anno l'effetto delle misure introdotte in precedenza. Nei prossimi giorni sarà perfezionata la messa a punto degli interventi che riteniamo necessario adottare per il prossimo trimestre, nell'intento di tutelare con continuità, in particolare in modo qualificato, i settori più esposti dell'economia e le fasce più vulnerabili della popolazione. Per quanto attiene all'opportunità di introdurre normativamente meccanismi che consentano di compensare gli effetti dell'inflazione con un proporzionale aumento del salario, ferma restando la necessità di tutelare il potere d'acquisto dei salari, ritengo rischioso prevedere istituti che potrebbero instaurare una spirale perversa tra inflazione e salari. Il Governo continuerà a tutelare le fasce più deboli utilizzando misure mirate e temporanee, che cercheranno di contemperare la sostenibilità della finanza pubblica con la necessità di mantenere un profilo di crescita sostenuta, prolungata e condivisa.

crea la ricchezza in questo Paese, consuma, produce e quindi è in grado di generare economia. In questo caso, i lavoratori, le lavoratrici in particolare e i pensionati sono quelli più penalizzati. Il dato è questo: una perdita di potere d'acquisto secca.

speriamo di avere, almeno in questa occasione, un po' di serietà sul tema, perché onestamente non guasterebbe, visti i tempi. L'Italia è rimasto l'unico Paese a non avere ancora ratificato la riforma del Trattato del meccanismo europeo di stabilità. La ratifica - è ormai chiarissimo a tutti - non imporrerebbe all'Italia di ricorrervi, mentre la sua mancata ratifica comporterebbe di fatto l'impossibilità di accedere a questo strumento per tutti i Paesi che vi hanno già provveduto. Nel Continente Nel Continente europeo - non so se questo Governo si sia reso conto di quello che sta accadendo - torna ad aleggiare anche il pericolo di una crisi nel sistema creditizio. Ora, è chiaro che si pone il problema di assicurare la piena operatività del meccanismo europeo di stabilità per rafforzare la capacità dell'Unione di fronteggiare eventuali situazioni di dissesto. Se l'ostruzionismo italiano perdurasse e fosse legato alla pretesa di modificare le finalità e le regole di funzionamento, questo contribuirebbe sicuramente all'isolamento politico dell'Italia nell'Unione europea, con conseguenze imprevedibili e certamente negative. Ministro, in queste ore il presidente del Consiglio Meloni è al Consiglio europeo e noi abbiamo uno straordinario bisogno di alleanze, di una capacità di ripresa del nostro Paese, di una capacità di dialogo e di autorevolezza dell'Italia in vari contesti. Il rischio reale è che il ritorno del presidente Meloni in Italia non porti grandi risultati rispetto a quello che sta accadendo ora nel Consiglio europeo. Mi chiedo come e quando il Governo deciderà in ordine alla presentazione di un disegno di legge per la ratifica del Trattato sul meccanismo europeo, perché penso che la questione sia profondamente legata anche a un ruolo più prestigioso e sicuramente più autorevole e di maggiore dialogo del nostro Paese con il resto dell'Europa. È un fatto che riguarda tutti noi, soprattutto in un momento in cui cui ricominciano a profilarsi sistemi e situazioni di difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti e che preoccupano anche i cittadini italiani.

ricordo agli onorevoli senatori interroganti come più volte in quest'Aula si sia tornati sul punto e, come ho già avuto modo di dire in Parlamento, che la risoluzione approvata il 30 novembre impegnava il Governo a non procedere alla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del MES con riferimento al quadro regolatorio europeo in evoluzione. Tengo a sottolineare che la riforma è stata concepita in un contesto diverso dall'attuale, che non teneva ancora conto degli *shock* determinati prima dalla pandemia e successivamente dalla crisi energetica correlata alla guerra tra tra Ucraina e Russia. Tali eventi hanno anche portato a un nuovo dibattito sulla *governance* europea e hanno mostrato quanto sia necessario procedere al completamento dell'architettura finanziaria europea, esattamente come richiamato nella risoluzione citata. L'Europa ha già compiuto progressi nell'integrazione economica, mirata non solo alla stabilità, ma anche alla crescita, attraverso il Next generation EU. Il tema della riforma del MES e, in particolare, il suo utilizzo come sostegno comune (*common backstop*) al fondo di risoluzione unico dovrebbe essere però inquadrato nell'ambito delle discussioni in corso sulla *capital markets union* e sull'unione bancaria. Sebbene quest'ultima in particolare sia ferma da troppo tempo per il veto di alcuni Paesi, con un comportamento che - usando i suoi termini - definirei a questo punto ostruzionistico, in realtà negli ultimi giorni ha in qualche modo rinnovato l'interesse a completare i tasselli mancanti di tale architettura finanziaria. È quindi nell'ambito di una complessiva e articolata riconfigurazione degli strumenti in grado di salvaguardare il mercato comune dalle turbolenze dei mercati finanziari che dovrà aver luogo il dibattito, anche parlamentare, sulla ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità.

Signor Ministro, devo confessarle che mi ero preparato una sorta di profezia per risponderle. Volevo dirle che, così come ci avevate detto che avreste smontato le accise, che avreste fatto il blocco navale, che avreste fatto la *flat tax*, che non avreste introdotto nuovi reati, eccetera, la mia profezia era che vi sareste rimangiati anche questa parola e che avreste ratificato il MES. Se ho capito bene la risposta sibillina che mi ha dato, io capisco così. E me ne compiaccio, signor Ministro, perché, guardi, il problema è che gli eventi a cui lei si è rifatto,

far parte di un consesso di Paesi nel quale si mantiene la parola e - me lo faccia anche dire - ci si difende pure, perché, ove mai ci fosse una crisi bancaria, signor Ministro, le nostre banche ovviamente ne soffrirebbero per prime. Abbiamo visto com'è andato il listino di borsa. Perché è stato proprio il listino di Milano a soffrire di più? Perché il nostro listino è pieno di titoli bancari. E allora, se non capiamo che questo è nell'interesse del Paese, ciò è molto preoccupante. La ragione, tra l'altro, è che voi siete un po' apprendisti stregoni, quelli che fanno gli incantesimi e non riescono poi a gestirne le conseguenze. La ragione per la quale non ratifichiamo il MES è la propaganda che avete fatto in questi anni, dicendo cose che non erano vere e confondendo per esempio le persone tra ratificare e prendere il MES; MES; adesso siete chiusi dentro una bolla e non sapete cosa fare. Vedrà però, signor Ministro, che sarà costretto a ratificare il MES, perché lo dicono il buon senso e le relazioni internazionali. Sono curioso di sentirlo, quando verrà qui a raccontarci che lo sta facendo.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, abbiamo avuto un Patto di stabilità e crescita che negli anni passati era molto più attento al tema della stabilità. Oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita. Questa dev'essere la nostra priorità. Le vecchie regole sarebbero oggi assolutamente irrealistiche e quelle nuove devono invece sostenere con efficacia i considerevoli investimenti pubblici necessari in questi anni in tutti i settori strategici, compresi l'ambiente, la difesa e la digitalizzazione. Il tempo dell'austerità è finito e il percorso di riequilibrio dei bilanci pubblici degli Stati maggiormente indebitati non dovrà sacrificare la dimensione dello sviluppo economico, non solo per evitare di colpire ulteriormente famiglie e imprese, ma anche perché la crescita economica stabile e duratura è l'unica vera garanzia di sostenibilità del del debito pubblico. Non sono parole mie, ma le sottoscriverei immediatamente, il che è piuttosto surreale, visto che sono parole della Presidente del Consiglio, rese in quest'Aula nella giornata del 21 marzo, quindi due giorni fa. Tuttavia, a parole così chiare rispetto al tema del debito, da un lato, e della necessaria crescita, dall'altro, dovrebbero conseguire fatti che, nella NADEF, nella legge di bilancio e in molte delle interlocuzioni che abbiamo avuto con il Governo, non abbiamo visto. Non voglio citare il superbonus, signor Ministro, ne abbiamo parlato pure troppo. Penso però a un piano di investimenti forte come il Piano transizione 4.0, che aveva aliquote di incentivo per credito d'imposta molto elevate e che ha visto, nel 2022, un più 14,3 di investimenti rispetto al 2021. Sarebbe stato necessario continuare su quella linea, quindi potenziare ulteriormente e non dimezzare le aliquote di transizione 4.0. Oggi l'Ufficio centrale di bilancio evidenzia che, nel nostro Paese, gli investimenti avranno un rallentamento pari al 2,7 per cento nel biennio, una minore propensione all'investimento da parte delle imprese, perché non sentono la fiducia nell'investimento. Ritengo invece che bisogni mettere in campo politiche economiche anticicliche, come abbiamo fatto in particolare nel Governo Conte II, abbiamo raggiunto dei risultati di crescita molto elevati, non soltanto di rimbalzo rispetto alla perdita di PIL nell'anno peggiore, quello del Covid-19, ma con misure che sostenevano una crescita duratura. Mi verrebbe da chiedervi cosa vi abbiano fatto le imprese italiane, che vengono penalizzate da una politica di bilancio che non tiene conto in nessun modo della necessità di favorire gli investimenti privati, proprio per poter sostenere la spesa pubblica e continuare a fare debito. Il problema della quantità di debito non c'è, infatti, se esso è sostenibile ed è sostenuto dalla crescita.

Di questa consapevolezza il Governo si fa carico, anche nell'ambito del difficile negoziato che, proprio in queste settimane, si sta svolgendo rispetto al nuovo patto di stabilità e crescita.

siamo al lavoro in un difficile negoziato, proprio per valorizzare la dimensione degli investimenti, pubblici e privati, in quella fase. Inoltre, credo che dobbiamo impegnarci moltissimo a sbloccare le risorse stanziate da tempo nei bilanci dello Stato, ma che in qualche modo non riescono a essere messe a terra. Cito, tra tutte, le risorse per i programmi di edilizia sanitaria: decine di miliardi che non riescono ad essere impiegati. Per quanto riguarda invece un altro aspetto che vorrei ricordare, una delle posizioni negoziali più forti che abbiamo assunto come Paese le misure per potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche alla luce dell'esperienza del cosiddetto Piano Juncker, che consentì di utilizzare risorse a leva per gli investimenti privati, con risultati più che positivi. Inoltre, presenterò presto al Consiglio dei ministri (auspicabilmente già la settimana prossima, in quanto mancano le ultime rifiniture), il disegno di legge collegato alla manovra pubblica, volto a favorire ed incentivare lo sviluppo del mercato dei capitali,

Abbiamo una domanda pubblica generata dal PNRR enorme. Il problema nostro è la capacità di rispondere con un'offerta adeguata, che colga quest'opportunità. Certamente lei, che ha fatto esperienze come me nel mondo delle imprese, capisce quanto sia importante. Faccio semplicemente un esempio: nel momento in cui c'è una rilevante domanda per infrastrutture pubbliche, occorre la capacità di un sistema di imprese e di opere pubbliche solido, in grado di intercettare queste gare e di realizzarle nei tempi più rapidi possibili.

siamo parti contrapposte in questa fase politica, ma perché mi aspettavo qualche elemento in più rispetto alle previsioni del DEF che state predisponendo e che penso vedremo È lì che si misurerà la volontà del Governo di sostenere la crescita. Oggi, anche dalle sue parole, vedo un po' di timidezza rispetto ai dati macroeconomici ed è evidente che

Credo che invece rispetto al tema europeo della *governance* e del Patto di stabilità e crescita che si lega, bisogni fare molta attenzione al tema degli aiuti di Stato, perché è evidente che concentrare la capacità dei singoli Stati membri di incentivare la crescita attraverso gli aiuti di Stato di Stato per noi, che abbiamo meno liquidità di altri Paesi più forti, può essere un vero problema. Credo allora che in quel negoziato la prima cosa da fare sia chiudere un pacchetto completo che tenga dentro anche le esigenze di Paesi quali la Germania in particolare e, in parte, la Francia, che non potranno aumentare il *range* di aiuto, perché non hanno la disponibilità finanziaria per farlo.

signor Ministro la transizione in chiave ecologica dell'economia, la transizione digitale, ambientale e sociale non possono rappresentare un incidente della storia. Sono e rappresentano una straordinaria opportunità per generare lavoro e nuovo sviluppo economico. Consideriamo lei e il suo Ministero cruciali per orientare al meglio gli investimenti, determinando azioni utili per spingere con moltiplicatori adeguati una buona e piena occupazione con una coerente gestione del debito. Noi riteniamo il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti, una proposta inadeguata, senza un'idea di come riordinare i *bonus* edilizi, una proposta che amplifica anziché risolvere i crediti cosiddetti incagliati; oltre 19 miliardi già maturati che mettono a rischio 115.000 cantieri, 32.000 imprese e 170.000 lavoratori. Mentre pensate di aver messo una pezza ai problemi del passato, si rischia una crisi sistemica dell'economia italiana. La carenza di liquidità spinge migliaia di imprese di costruzioni verso procedure fallimentari. Quando si perde un'impresa, si riduce l'occupazione, crescono tensioni sociali ed il Paese perde un'idea e un progetto dello sviluppo economico difficilmente ricostruibili in tempi brevi. Signor Ministro, sono le stesse imprese che poi dovrebbero operare per dare piena attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo consapevoli che una misura come il 110 fosse utile per far ripartire il Paese dopo una pandemia, per rilanciare gli investimenti e garantire una crescita economica più elevata, ma per i costi elevati non poteva essere una misura strutturale. Nello stesso tempo, le importanti azioni in atto per contrastare e sradicare l'illegalità rendono certamente le istituzioni più credibili e più solide, ma non possono determinare il blocco totale delle cessioni dei crediti, a maggior ragione nei confronti di quelle imprese e quelle famiglie che, rispettando le norme dello Stato, hanno operato nella legalità e si ritrovano cantieri bloccati, contenziosi immediati con la pubblica amministrazione e del sistema del credito, ammortizzatori sociali al posto del lavoro. Sono famiglie che si sono affidate ad un progetto delle nostre Istituzioni. Signor Ministro, per governare un grande Paese manifatturiero non è sufficiente fare opposizione al passato; se non si introducono misure urgenti per affrontare il presente, non si coglie il futuro. Agite in fretta, il tempo sta passando. Noi abbiamo avanzato diverse proposte, a cominciare dall'utilizzo degli F24 a compensazione dei cosiddetti crediti maturati. Abbiamo avviato iniziative importanti e proposte anche per coinvolgere le nostre partecipate pubbliche. Non possiamo giocarci l'esigenza di rigenerare il nostro patrimonio edilizio, la casa, per migliorare la qualità dell'aria e garantire la sicurezza statica del nostro patrimonio residenziale e produttivo. Rigenerare, rinnovare e riqualificare le nostre città è un'esigenza per evitare un insostenibile consumo di suolo. Occorrono misure urgenti. Non abbiamo quarantotto mesi per dare attuazione ai nuovi decreti, ma avete pochi giorni per sbloccare, dico io, i crediti bloccati e salvaguardare l'occupazione e lo sviluppo economico delle nostre imprese e delle nostre famiglie che hanno agito nella legalità.

penso che non vada negato che il superbonus abbia rappresentato, in una precisa fase storica, un impulso alla ripresa e al lavoro.

per stimolare interventi che, a conti fatti, vanno a interessare meno del 5 per cento del patrimonio immobiliare esistente. Per noi il successo è riuscire a fare molto con poco, non riuscire a fare poco con molto. La decisione che il Governo ha preso il 16 febbraio prevede comunque la disciplina transitoria, che consentirà di continuare a esercitare le opzioni di sconto e cessione per tutti gli interventi per i quali risultano già presentate le richieste di titolo edilizio abilitativo, proprio per tutelare il principio di legittimo affidamento di chi, pur non essendo magari ancora partito con i lavori, si trovava la data di blocco già in una fase avanzata di progettazione degli interventi. I cosiddetti esodati esistevano già a quella data, non li ha certo creati il decreto-legge adottato da questo Governo, ma i decreti assunti in precedenza. Il Governo comunque ha adottato il decreto-legge che cerca di dare certezze per quanto riguarda questi crediti ai fini degli acquisti. Nel corso del dibattito in Commissione alla Camera sono già stati approvati emendamenti tesi a favorire in particolare la continuazione delle attività per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, le ONLUS e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Continuiamo a lavorare anche dietro le quinte, consapevoli che per chi in questa trappola ci è già caduto e si ritrova a lavorare con crediti incagliati, nati non in relazione al nostro decreto, una soluzione vada trovata e ci impegneremo fino all'ultimo minuto utile per farlo, perché si tratta di famiglie ed imprese che in buona fede hanno creduto ai fuorvianti messaggi iniziali della gratuità per tutti e senza costi per nessuno. Infine, merita un cenno la sollecitazione degli onorevole interroganti circa la necessità di immaginare quello che potrà essere il futuro. Fra tante incertezze, vi sono due certezze: la prima è che una nuova stagione di *bonus* al 110 per cento per tutti, ricchi e poveri, prime e seconde case, al mare o in montagna, non è all'orizzonte. La seconda è che un dosaggio mirato di percentuali di detrazioni spettanti e di perimetrazione accurato di tipologie di interventi per i quali consentire ancora, in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive, quali il disagio economico e sociale, sconti e cessioni, costituirà un'ipotesi di futuro sostenibile. Concludo dicendo che ritengo ragionevole, al di là della prudenza che mi contraddistingue, proprio grazie al lavoro, anche oscuro e non pubblico, che ha fatto il Governo in queste settimane, che nei prossimi giorni vi saranno notizie positive. Per tutti questi esodati da provvedimenti di Governi precedenti, una soluzione sarà trovata. colleghi, ho troppa stima nei confronti del Ministro e del Ministero che rappresenta per dover ricordare che insieme abbiamo governato il Paese durante l'esperienza del Governo Draghi e insieme abbiamo anche tentato di affrontare questo tema. Credo che la questione che abbiamo posto non si risolva nel fare opposizione al passato, ma si risolva se affrontiamo il presente e il futuro, in modo particolare sul tema delicato che abbiamo posto. Siamo infatti in presenza di migliaia di imprese a rischio di liquidità liquidità e probabilmente molte di queste azioni, che hanno coinvolto famiglie e imprese, si sono svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti. Pertanto, in un Paese in cui giustamente, secondo me tardivamente, insieme, e dico così perché eravamo insieme al Governo l'esperienza del Governo Draghi - abbiamo avviato le azioni utili e necessarie, che dovevano essere avviate prima, per sradicare l'illegalità e per non confondere la legalità con l'illegalità, credo che con altrettanta forza e determinazione dobbiamo dare una risposta a quelle imprese e a quelle famiglie che, agendo nella legalità, si sono fidate dello Stato. hanno fatto investimenti importanti nelle imprese, per riqualificare il comparto delle costruzioni, verso la rigenerazione, che è un'operazione economica e sociale indispensabile, se guardiamo al futuro delle costruzioni nel nostro Paese, che sarà sempre di più orientato alla rigenerazione urbana rispetto al consumo di suolo. Se temporeggiamo e perdiamo tempo nelle accuse al passato, rischiamo di perdere di vista un'emergenza. Penso sia necessaria una norma quadro per riordinare i *bonus* edilizi, per dare una prospettiva al settore e per farlo anche con finanza europea, perché le direttive europee vanno accompagnate dalle risorse, per costruire le condizioni nel Paese per consumare meno energia, per garantire maggiore tenuta statica ai nostri fabbricati e per evitare il consumo di suolo, che oggi è insostenibile, per le dotazioni e la qualità della vita, ma anche per dare un'idea di città in cui gli *standard* pubblici tornino a favorire coesione e relazioni tra le persone. Ci stiamo cioè giocando il comparto produttivo più importante per abitare il presente e il futuro. Facciamo in fretta ed è per questo che non mi convincono le impostazioni del decreto, perché avrei messo, a fianco del decreto, una norma quadro per dare un riordino complessivo a tutti i *bonus* in edilizia, per dare certezza al comparto e per sbloccare i crediti che legittimamente le imprese hanno adottato nel rapporto con il sistema del credito. Pertanto voglio vedere le condizioni alle quali lei fa riferimento... delle notizie che ci ha dato, dobbiamo vedere nella coerenza e nella concretezza i provvedimenti che ha annunciato. Per ora non siamo soddisfatti, perché continuano ad essere a rischio famiglie e imprese italiane.

il nostro quesito riguarda i congedi parentali, che come lei sa benissimo sono un dispositivo sociale in continua evoluzione, come è ovvio che sia, trattandosi di una contromisura che viene assunta per favorire la soluzione di bisogni delle famiglie che cambiano nel tempo. Nonostante quindi la normativa vigente preveda che i congedi possano essere utilizzati da entrambi i genitori e che la coppia venga premiata con un mese aggiuntivo se il padre prende almeno tre mesi di congedo, i dati ci dicono che solo il 26,9 per cento degli uomini ne usufruisce, a fronte del 68,6 per cento Allo stesso tempo si registra una forte divaricazione tra il settore pubblico, dove il 34,1 per cento degli uomini usufruisce dei congedi, e quello privato, dove la percentuale scende al 19,8 per cento. In tale contesto le ripercussioni sull'occupazione femminile sono purtroppo inevitabili.

La fruizione del congedo comporta una notevole perdita di reddito per la famiglia e il primo percettore di reddito, generalmente il padre, è in grado di esercitare il proprio diritto al congedo solo se quest'ultimo è sufficientemente retribuito, come bene dimostrano le esperienze di successo di altri Paesi europei, non solo del Nord Europa, ma anche, ultimamente, della Spagna. Proprio la scorsa settimana, rispondendo a un'interrogazione alla Camera, la presidente Meloni ha confermato che il sostegno alle madri lavoratrici è una priorità assoluta dell'Esecutivo. Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se lei non ritenga che il congedo parentale retribuito all'80 per cento - come attualmente avviene solo per il primo mese per più tempo sia la soluzione più efficace per dare effettivo sostegno alle madri lavoratrici e se si tratti di una misura che in concreto si può impegnare a realizzare nell'ambito del suo Dicastero. La ringrazio, signora Ministra.

ringrazio gli interroganti per l'importante tema sollevato, perché la conciliazione tra lavoro e vita privata, con particolare riguardo alla cura dei figli, è un pilastro delle politiche familiari e demografiche. Tutte le rilevazioni, anche in tema di natalità, sottolineano l'importanza della flessibilità oraria e della disponibilità di congedi familiari. Attualmente il congedo parentale spetta ai genitori lavoratori entro i primi dodici anni di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. I congedi possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. Va sottolineato che, in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto spetta alle stesse condizioni per ogni bambino. La legge di bilancio per il 2023 ha introdotto un'importante novità che dispone, per massimo un mese e fino al sesto anno del bambino, l'elevazione dell'indennità dal 30 all'80 per cento della retribuzione, nel senso auspicato dall'interrogante. Tale incremento è peraltro anche coerente con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, che prevede sia un aumento dell'indennità sia l'aumento dei giorni di congedo parentale per i padri, in continuità con il già previsto aumento a dieci giorni. I limitati margini finanziari hanno permesso una riforma parziale dell'istituto, che andrebbe sicuramente potenziato nella direzione già intrapresa da questo Governo, anche valutando un utilizzo flessibile della percentuale della retribuzione nel periodo di congedo. I congedi parentali rientrano tra l'altro in una più ampia strategia di valorizzazione della maternità e della paternità in ambito produttivo. Abbiamo lanciato infatti anche un codice di autodisciplina per le imprese in tema di maternità che, in dialogo con le parti sociali e datoriali, promuova l'adattamento dei tempi e dei modi di lavoro. Tra le proposte c'è la possibilità di congedi e aspettative più lunghi rispetto alla legge e al contratto collettivo, integrabili economicamente tra l'80 e il 100 per cento, in ottica collaborativa tra aziende e dipendenti,

sia nei principi generali, cui dovranno ispirarsi le politiche di incentivazione, sia come criterio specifico per la redazione del codice degli incentivi. la ringrazio per queste sue parole; ho apprezzato molto il fatto che lei dica che si tratta di un dispositivo che dovrebbe essere potenziato, perché questo va nella direzione della nostra interrogazione. che qualcosa si muova. Tutte le altre considerazioni che lei ha fatto sicuramente depongono a favore di un'evoluzione delle modalità di gestione delle lavoratrici nell'ambito del nostro sistema economico, ragion per cui mi considero almeno parzialmente soddisfatto, nell'attesa che si muova qualcosa nella

pari opportunità* - Premesso che: non è vero, come da qualcuno sostenuto, che i bambini che vivono con coppie dello stesso sesso, se nati all'estero, non possono essere iscritti all'anagrafe se vengono in Italia, e quindi non abbiano dei diritti,

particolare: se due uomini all'estero ricorrono alla pratica dell'utero in affitto e sono riconosciuti entrambi padri di un bambino, quando vengono in Italia sarà padre quello il cui cognome compare nel certificato di nascita del piccolo, e solitamente coincide con il padre biologico; se due donne all'estero ricorrono alla fecondazione assistita e sono riconosciute entrambe madri di un bambino, quando vengono in Italia sarà riconosciuta madre quella che ha partorito; in ogni caso il bambino viene registrato in Italia senza problemi all'anagrafe, con un solo genitore. Ci si chiede quali sarebbero i diritti negati: il bambino avrà gli stessi diritti di qualsiasi altro bambino con un genitore; il problema delle trascrizioni sorge perché le coppie di uomini o donne che hanno avuto figli ricorrendo alla pratica dell'utero in affitto o alla fecondazione assistita eterologa, all'estero, vorrebbero essere riconosciuti anche in Italia entrambi padri o madri. Vogliono cioè che sia trascritto un atto che in Italia non esiste.

quali siano le politiche del Governo in materia, con particolare riguardo alle attività di competenza del suo Ministero che - mi rendo conto - non ha la competenza su tutti gli aspetti giuridici, ma è un Ministero importante e la ringrazio per l'azione che sta svolgendo su questi temi.

Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti perché il tema sollevato è stato oggetto in questi giorni di importanti dibattiti nel Paese, quindi ha assunto una centralità a cui è bene dare risposta. Come giustamente ricorda l'interrogante, non sono in discussione i diritti dei bambini in Italia, anche se nati all'estero con pratiche che sono reato nel nostro Paese, come ad esempio la maternità surrogata (o utero in affitto), vietata dalla legge n. 40 del 2004, attualmente ancora vigente. Ricordiamo infatti che nel caso di un atto di nascita prodotto all'estero in cui risultino genitori due padri, la trascrizione in Italia prevede quella del solo padre biologico. Una volta riconosciuto il genitore biologicamente legato a sé, il piccolo potrà godere immediatamente di tutti i diritti, dall'assistenza sanitaria all'istruzione, come già accade ad esempio ai bambini non riconosciuti dal padre e cresciuti da madri cosiddette *single.* È quindi importante ribadire che non c'è nessuna discriminazione nei confronti dei bambini e lo dico proprio perché lei si è riferito alle competenze del mio Ministero, che sono sicuramente contro le discriminazioni. Questa discriminazione sarebbe del resto inaccettabile. Permane la condanna dell'utero in affitto stabilita dalla legge n. 40 del 2004 e ribadita più volte da diverse sentenze della Corte costituzionale. Recentemente anche la Corte di cassazione, il 30 dicembre 2022, a sezioni unite, con la sentenza n. 38162 ha affermato con chiarezza che tale pratica: «[...] offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale.». Nella stessa sentenza la Corte di cassazione ha poi indicato che: «L'automatismo del riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione sulla base del contratto di maternità surrogata e degli atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante da questo contratto non è funzionale alla realizzazione del migliore interesse del minore, attuando semmai quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi.». La Corte ha quindi escluso ogni automatismo nella trascrizione degli atti di nascita prodotti all'estero a seguito di procedure di utero in affitto, sottolineando come la trascrizione automatica non sia in funzione dei diritti del minore, ma di quelli dell'adulto. Richiamando precedenti sentenze in merito sia della stessa Cassazione che della Corte costituzionale, la pronuncia dello scorso dicembre individua quindi nell'adozione in casi particolari previsti dalla legge n. 184 del 1983 il percorso da seguire per eventualmente assicurare il rapporto genitoriale del minore con il *partner* del genitore biologico. biologico. Nei propri atti, il Governo è dunque tenuto al rispetto del quadro normativo che ho illustrato, sul quale poi è facoltà del legislatore eventualmente intervenire.

presente nel nostro Paese, vengono rispettati e garantiti: questo viene ribadito, perché si fa una propaganda mistificante su questa materia. Dopodiché lei ha detto una cosa importante, parlando "del figlio ad ogni costo" e lo dico davanti a un Ministro che deve occuparsi di famiglia e favorire politiche di natalità. Il nostro Paese ha perso 400.000 abitanti in tre anni e ha un problema di tutela della famiglia e della natalità. Non si può però andare oltre le barriere del diritto naturale, per cui il figlio ad ogni costo è una forma di egoismo, che porta alla compravendita di ovociti, alla scelta della donna in cui poi impiantarli, perché le esigenze sono diverse, con uno spirito talvolta quasi razzista nelle scelte che vediamo illustrate in fiere internazionali, che fanno una sorta di tratta delle persone. Ben venga, quindi, un'ulteriore legge - anch'io ne ho presentata una di questo tenore al Senato che metta al bando queste attività fatte all'estero da italiani: non vogliamo legiferare negli altri Paesi, ma sanzionare i comportamenti di italiani che ricorressero alla pratica dell'utero in affitto altrove. La mercificazione del corpo delle donne e la compravendita di bambini sono attività spregevoli. I diritti dei bambini sono invece una priorità sacrosanta e ci aspettiamo un coro unanime, quando si discuteranno alla Camera - che ha già incardinato il le norme contro l'utero in affitto. Aspettiamo tutti al banco di prova *(Applausi)*, perché esistono anche i diritti delle donne e i diritti dei bambini a non essere comprati e venduti. Andiamo avanti per tutelare i bambini, le famiglie e anche il diritto naturale.

Signor Presidente, signor Ministro, da novembre 2022 in Iran si susseguono casi di avvelenamenti all'interno delle scuole del Paese rivolti a studentesse di tutte le età. di ragazze nel corso dei mesi sono state costrette al ricovero con chiari sintomi di intossicazione grave per via respiratoria. Nonostante le famiglie delle studentesse vittime degli attacchi abbiano sollecitato le autorità su quanto stesse accadendo tramite *sit-in* e manifestazioni, inizialmente le istituzioni le istituzioni locali e nazionali hanno deliberatamente liquidato le segnalazioni. Dopo migliaia di casi, che si sono moltiplicati in tutti i grandi centri urbani del Paese, le autorità, tramite le parole del Vice Ministro della salute, hanno confermato che tali episodi erano realmente degli avvelenamenti intenzionali che, come oramai come oramai risulta chiaro, hanno come obiettivo immediato quello di impedire alle studentesse di frequentare le scuole, ma come obiettivo politico quello di vietare l'educazione all'intero genere femminile. Episodi analoghi di avvelenamento avvennero anche anni fa in Afghanistan e avevano il medesimo obiettivo, che oggi vediamo esemplificato con il divieto totale di accesso all'educazione per le donne nel Paese guidato dai talebani. Concludendo, ricordo che lo scorso 16 marzo il Parlamento europeo ha votato ad ampia maggioranza una risoluzione che, tra i vari impegni, esorta il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a dare il via a un'indagine indipendente sugli avvelenamenti delle studentesse. Ricordo inoltre, come abbiamo fatto ieri in Aula, che da mesi la società civile le donne in special modo protestano per chiedere diritti e libertà a un regime totalitario e oppressivo. Si chiede pertanto di sapere, al fine di chiarire i gravi episodi di avvelenamento esposti in premessa, che rischiano di indebolire ulteriormente la società civile iraniana, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, intraprendere, insieme ai *partner* europei, per dare seguito alla volontà di incaricare una missione indipendente per accertare i fatti.

quello che stava accadendo, chiedendo l'immediata cessazione della repressione. Come sapete, ho per questo convocato l'ambasciatore iraniano prima ancora che fosse accreditato; ambasciatore poi autorevolmente richiamato dallo stesso Presidente della Repubblica. Noi continuiamo ad agire insieme ai *partner* dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. I primi casi di avvelenamento risalgono a novembre scorso, ma solo ora, dopo pressioni mediatiche, le autorità iraniane hanno voluto mostrare di essersi attivate e di aver individuato i responsabili: hanno quindi annunciato l'arresto di circa cento persone accusate di essere legate a gruppi ostili. Le autorità iraniane attribuiscono la responsabilità dei fatti a entità esterne, gruppi terroristici vicini all'ideologia talebana e ai cosiddetti Mojahedin del Popolo, che Teheran considera anti-regime. L'opposizione fa invece riferimento a responsabilità interne, nate dalla volontà di punire la partecipazione alle manifestazioni di protesta. Ciò giustificherebbe la debole risposta delle autorità, i lenti tempi di reazione, gli scarsi mezzi investigativi che sono stati impiegati. La vicenda rischia di avere di avere delle ripercussioni molto forti sul funzionamento delle scuole straniere presenti in Iran. Anche la scuola italiana di Teheran ha rafforzato i dispositivi di sicurezza. L'Italia mantiene altissima l'attenzione sulla questione e continueremo in particolare ad adoperarci perché, sia a livello bilaterale che multilaterale, messaggi chiari e improntati alla massima fermezza siano rivolti alle autorità

ragazze dopo le proteste iniziate il 16 settembre. Si raccoglieranno evidenze utili per futuri procedimenti avviati da corti o tribunali internazionali e regionali. La missione, composta da esperti indipendenti, è chiamata a riferire al Consiglio in occasione della prossima sessione di giugno a Ginevra. Tutti presteremo massima attenzione alle risultanze del rapporto della missione di accertamento dei fatti. In sede In sede di dibattito, l'Italia ribadirà la necessità di accertare le responsabilità degli episodi di avvelenamento. Sosterremo inoltre il rafforzamento della collaborazione tra la missione conoscitiva internazionale e il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, anche sui casi di avvelenamento. Non mancheremo, infine, di ribadire la nostra attenzione anche in occasione delle riunioni di coordinamento europeo, che accompagnano la sessione di lavoro del Consiglio dei diritti umani. Fermezza e vigilanza sulle violazioni dei diritti umani, in modo particolare delle donne, continueranno a rappresentare una priorità per questo Governo. che, come Gruppo parlamentare, il lavoro svolto assieme ai colleghi del Parlamento europeo dimostri l'impegno che portiamo avanti proprio per far sì che l'attenzione su quanto sta accadendo in Iran sia mantenuta. convinti che la lotta della società civile iraniana e la lotta delle donne iraniane contro una teocrazia dai tratti palesemente reazionari debba debba continuare a trovare spazio nel dibattito pubblico e politico. Non possiamo permetterci di abbandonare milioni di donne e un popolo che sta semplicemente chiedendo più diritti e più dignità.

*(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, prendo la parola per illustrare questa interrogazione che ho depositato con altri colleghi del Gruppo di Fratelli d'Italia proprio sulla questione tunisina, tunisina, che è stata affrontata su richiesta italiana lunedì scorso, il 20 marzo, al Consiglio degli affari esteri dell'Unione europea, dove l'Italia si è fatta promotrice di una richiesta di aiuto rispetto a una Nazione in enorme difficoltà.

È una Nazione che quindi riesce con enorme difficoltà a trovare le risorse per portare avanti la propria azione di Governo, stretta in una crisi economica in cui sicuramente da un lato l'uscita dalla pandemia, dall'altro i riflessi della crisi russo-ucraina hanno una loro incidenza ma non sono esclusivi. che riguarda la Tunisia non è fondamentale da un punto di vista italiano solo per la vicenda dei flussi migratori (purtroppo le cronache delle ultime ore ci continuano ad addolorare); non è fondamentale solo per l'approvvigionamento energetico (sappiamo che l'Italia ha negli ultimi anni aumentato di gran lunga la possibilità di approvvigionamento soprattutto di gas dalla Tunisia), ma è fondamentale anche da un punto di vista commerciale, se è vero come è vero che nel 2022 per la prima volta l'Italia è diventato il primo *partner* commerciale della Tunisia superando la Francia. È chiaro, quindi, che abbiamo un interesse strategico nazionale non solo per le quasi mille imprese a capitale italiano che operano sul territorio tunisino, ma proprio per una stabilizzazione di quell'area che risulta assolutamente fondamentale per curare il nostro interesse. La domanda che formuliamo con questa interrogazione, pertanto, è quali siano quali saranno le iniziative che il Governo italiano o l'Unione europea intende porre in essere per cercare di alleviare una situazione che è sull'orlo della drammaticità. *(Applausi)*.

l'attenzione del Governo per la crisi economico-finanziaria della Tunisia è massima, in considerazione non soltanto delle ripercussioni migratorie, ma soprattutto di quelle politiche nell'intera Insieme al Presidente del Consiglio, ma anche con il ministro Giorgetti, stiamo sensibilizzando tutti i *partner* europei e internazionali sull'urgenza di garantire adeguato sostegno alla alla Tunisia. È in programma anche oggi, nel tardo pomeriggio, una nuova telefonata con la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, per discutere proprio di questo. L'accordo con il Fondo monetario per un credito di 1,9 miliardi di dollari è cruciale nell'immediato e in prospettiva futura. L'intervento offrirebbe la base per ulteriori programmi di sostegno sul piano bilaterale e multilaterale. Allo stesso tempo, incoraggiamo le autorità tunisine a proseguire il programma di riforme economiche. Anche nel Consiglio affari esteri di lunedì scorso a Bruxelles, che ha affrontato - su mia richiesta - il punto della crisi tunisina, è stata sottolineata l'importanza che l'Unione europea consideri la Tunisia una priorità e agisca rapidamente. Il suo collasso colpirebbe innanzitutto l'Italia, ma con ripercussioni immediate sul resto d'Europa. I flussi migratori crescerebbero esponenzialmente e le conquiste della democrazia tunisina degli ultimi anni Piangiamo anche noi le vittime del naufragio di qualche ora fa, che ha visto morire molti cittadini della Costa d'Avorio. Per questo a Bruxelles ho insistito sulla necessità che l'Europa si mostri al fianco del popolo tunisino in un momento di profonda difficoltà. Su questo nostro impulso, l'Unione europea ha ribadito l'impegno ad assistere Tunisi sotto il profilo economico-finanziario e nel campo del contrasto alla immigrazione irregolare e ha attivato una missione del commissario Gentiloni già nei prossimi giorni; missione alla quale seguirà quella dei Ministri degli esteri di Portogallo e Belgio in nome e rappresentanza del Consiglio affari esteri. L'Italia sta facendo naturalmente la propria parte. Siamo pronti a considerare ulteriori interventi per favorire la crescita e quindi la stabilità della Tunisia. Abbiamo recentemente approvato il rifinanziamento di un credito d'aiuto del valore di 55 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese tunisine e il 65 per cento sarà destinato ad acquisti di beni e servizi italiani. Abbiamo previsto un sostegno al bilancio tunisino. Si tratta di 50 milioni di euro a credito, cui sono associati 3 milioni a dono. L'intero ammontare è destinato a promuovere efficienza energetica ed energie rinnovabili. Uno sforzo coerente con l'impegno italiano a favore dell'elettrodotto Elmed, progetto strategico per collegare le due sponde del Mediterraneo, che si inquadra nella volontà del nostro Governo di fare dell'Italia un *hub* energetico. La Tunisia è per noi un Paese prioritario. I contatti che intrattengo con il collega Ammar, ministro degli esteri, sono continui, anche sulla scia della mia missione a Tunisi a gennaio con il titolare del Viminale, il ministro Piantedosi; missione cui abbiamo voluto dare seguiti concreti, valutando nuovi progetti di cooperazione, anche con riguardo a possibili iniziative in temi di premialità per i rimpatri e di sicurezza alimentare. Il Governo continua a seguire da vicino gli sviluppi della situazione in Tunisia. Ribadiamo vicinanza e amicizia al popolo tunisino, per favorire lo sviluppo e la stabilità del Paese, evitarne il tracollo e le sue ripercussioni migratorie e politiche e tutelarne la democrazia.

lascia intravedere una visione chiara del Governo e del suo Ministero rispetto a una linea di politica estera che, se mediaticamente è comprensibilmente accentrata sulla vicenda russo-ucraina, è altresì vero che presenta una serie di scenari

quasi di confine e che non influisce sulle politiche e sulla crescita degli Stati europei, come invece in realtà è. Penso non solo alla vicenda tunisina, di cui lei ovviamente nella risposta ha dato il percorso, illustrando quello che si cercherà di fare per

Tale ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite e quest'anno il tema riguarda il legame tra l'acqua e i cambiamenti climatici; quindi il messaggio è quello di ridurre gli sprechi e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Stiamo vivendo un allarme mondiale e il fatto che la siccità si stia protraendo da oltre due anni ci induce a riflettere sulle nostre responsabilità. Come autorevolmente scrive il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano e uno tra i maggiori esperti e studiosi (autore di diversi libri) in tema di suolo e di questioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche, se non piove è a causa dei cambiamenti climatici, che a loro volta sono conseguenza del nostro modo di abitare la terra e di non considerare che le risorse sono scarse. scarse. Occorre mettere in relazione tra loro le risorse, considerandole interdipendenti e facenti parte di un unico grande ecosistema (l'acqua con il suolo, il suolo con le piante, le piante con l'aria, l'aria con il suolo), e comprendere che danneggiare una parte significa finire per danneggiare le altre. Il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti, come ricordato il 21 aprile scorso nella risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo. Quindi, se manca l'acqua è anche perché trascuriamo i suoli che potrebbero trattenerla. Perché consumiamo il suolo, alterando il ciclo delle acque, con tutti i danni che ne conseguono? Siamo fissati su agricolture intensive, non più ammissibili e perché promuoviamo una dieta alimentare super idroesigente. Occorre, dunque, avviare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare altrettanto. Urbanizzare un prato significa rinunciare a far infiltrare un quantitativo di acqua di pioggia fino a quattro o cinque volte di meno e questo aggrava gli effetti della siccità. Lo deve sapere l'urbanista e lo deve sapere il sindaco quando approva un piano urbanistico con nuove e vecchie urbanizzazioni. Il 50 per cento della pioggia si infiltra solo se incontra superfici a prato o a bosco. Se queste diminuiscono, specie in pianura, è un grave problema. La metà dell'acqua che si infiltra scende in falda e l'altra metà rimane nei primi centimetri di suolo, che dobbiamo pensare come ad una grande cisterna, che accumula acqua preziosa per restituirla poco alla volta alle piante, quindi, anche quando non piove, e soprattutto quando non piove. Tutta l'acqua che rimane in campo è acqua preziosa che non perdiamo. Se, invece, cementifichiamo, le poche acque di pioggia scorreranno via velocemente, rischiando pure di fare gravi danni se la pioggia sarà intensa e breve. Un suolo non urbanizzato può trattenere fino a 3,8 milioni di litri